avverto che la prevista informativa del Ministro dell'interno sulla questione dei flussi migratori provenienti dal Nord Africa avrà luogo nella seduta antimeridiana di domani, con inizio alle ore 11. I Gruppi avranno a disposizione dieci minuti ciascuno per i propri interventi. Il Gruppo Misto

sono trascorsi due anni dal gravissimo sisma che ha colpito, nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 aprile 2009, la città dell'Aquila e la sua provincia. Quella mattina d'aprile l'Italia intera sostò attonita e commossa di fronte alle terribili distruzioni provocate dalla violenza del terremoto, che in pochi secondi ha mietuto più di trecento vittime, devastato migliaia di case e sfigurato tanti preziosi segni di una identità civile, artistica e spirituale di antichissima e nobile origine. Il popolo d'Abruzzo, così duramente colpito da quella immane tragedia, ha mostrato a tutti noi e al mondo intero una tempra eccezionale, grazie alla quale ha saputo reagire ai lutti e alle distruzioni ed iniziare a ricostruire il tessuto sociale, civile e produttivo sconvolto dalla violenza della natura. Molti sforzi sono stati compiuti, in questi due anni, per restituire una casa a migliaia di famiglie, rilanciare le attività economiche, ricostituire il tessuto civile e culturale - dalle istituzioni locali all'università - e recuperare gli ingentissimi danni al patrimonio artistico. Come ho già affermato nel messaggio inviato al prefetto dell'Aquila, il profondo dolore di quei giorni non deve offuscare il grande lavoro di quanti - istituzioni e privati cittadini - hanno saputo operare per il bene comune. È allora ancor più necessario continuare ad investire le nostre migliori energie nell'obiettivo di tornare a far risplendere quei centri storici che, all'Aquila come nelle altre comunità della sua provincia, costituiscono il fulcro del nostro modello di convivenza civile: soltanto allora potrà dirsi veramente compiuta l'opera di ricostruzione. Voglio esprimere ancora una volta, a nome di tutta l'Assemblea, profonda vicinanza alle popolazioni colpite da quella immane tragedia, ed immutata gratitudine verso tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato al soccorso e stanno ancora collaborando alla ricostruzione: un impegno corale che costituisce - lo ribadisco - l'espressione più autentica della profonda coesione del nostro Paese. In questo spirito di solidarietà umana ed istituzionale, invito allora tutti i colleghi ad osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento, in memoria delle 309 vittime del terremoto.

Presidente, colleghi, sono trascorsi due anni dal terribile terremoto che, nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 aprile 2009, ha colpito la città dell'Aquila e la sua provincia. Quei 309 rintocchi di campana sono nel cuore di tutti noi. Il nostro Paese ha dimostrato in questa occasione un encomiabile senso di responsabilità e solidarietà e, accanto a coloro che si sono generosamente impegnati in prima persona nel soccorso e nella ricostruzione, altissimo è stato il numero di quelli che, dall'Italia e dall'estero, hanno dato vita ad una straordinaria gara di solidarietà per sostenere gli sforzi dei soccorritori e lenire il dolore delle vittime. A due anni dall'immane tragedia che ha colpito la città dell'Aquila, il suo circondario e l'Abruzzo intero, ci corre l'obbligo, prima morale, poi politico ed istituzionale, di gettare uno sguardo sul passato recente e di proiettare la nostra attenzione verso il futuro, perché il futuro degli aquilani non è di corto respiro ma riguarda certamente il prossimo decennio. Le commemorazioni come questa sono utili e valide se tendono verso la verità e se costituiscono un insegnamento per guidare le vicende a venire. Per cui non faremmo cosa utile se in questo momento non guardassimo allo scenario di due anni fa: una tragedia immane per le vittime, le sofferenze fisiche e morali e i danni materiali, in una città storica con un enorme patrimonio culturale e artistico, con grandi potenzialità turistiche da conservare gelosamente e valorizzare come fondamento di memorie, tradizioni e valori, ma anche di progresso e sviluppo economico. Per non parlare della sua università, vero motore di cultura e di ricchezza, e delle istituzioni pubbliche, tutte rase al suolo o comunque rese inagibili. Solo partendo da questo scenario possiamo comprendere come si sia parlato e si continui a parlare di un vero e proprio miracolo aquilano. In prima linea, come certamente era suo dovere istituzionale, c'è stato il Presidente del Consiglio con l'intero Governo, ma anche tanti rappresentanti politici ed istituzionali dell'una e dell'altra parte, a partire dal sindaco dell'Aquila e dai sindaci dei tanti Comuni colpiti dal terremoto, sia dell'aquilano che del pescarese e del teramano. Ma la risposta fu resa possibile soprattutto dall'organizzazione della Protezione civile, che tutti ci invidiano: un'organizzazione che mette insieme il meglio dei nostri organismi pubblici ma anche il meglio dell'impegno civile e sociale, rappresentato da quei tanti volontari che ci rendono orgogliosi di chiamarci italiani. Non vogliamo, Presidente, assolvere, ma neanche condannare nessuno. Vogliamo solo ricordare che fra il facile ottimismo e il catastrofismo esiste una terza via, quella della razionalità, e questa ci induce a ripartire dal ricordo della maturità, responsabilità e dignità con cui gli abruzzesi hanno sopportato il terremoto, hanno pianto sui loro morti e stanno affrontando le disastrose conseguenze,

riguarda i sopravvissuti, queste vittime invisibili che hanno diritto al futuro e giustamente non si abituano ad una città che non esiste più e che in due anni non poteva ragionevolmente pensarsi potesse tornare a essere quella che era. era. Si devono infatti ricostruire non solo le case, le chiese, i luoghi di incontro e socializzazione, ma la sua identità e persino i tempi e i luoghi del quotidiano, quei tempi che rappresentano, per i più anziani, un patrimonio sottratto per sempre e, per i più giovani, un patrimonio che potranno conoscere solo per narrazione, un patrimonio materiale e immateriale che si ricostruirà nel tempo con la forza e la volontà degli abruzzesi, ma anche con la rinuncia da parte di tutti noi agli egoismi localistici. Investire nel recupero rapido della dimensione urbana, storica e identitaria strappata drammaticamente agli aquilani non dipende solo dal Governo. Siamo in un momento di crisi: dobbiamo fare delle scelte, dobbiamo agire con saggezza e razionalità e limitare le richieste. Avremo forse qualche voto in meno nelle nostre circoscrizioni, ma avremo il vanto di aver voluto recuperare un patrimonio artistico e umano che appartiene non solo agli abruzzesi

Signor Presidente, la ringrazio per le parole che lei ha rivolto all'Aula. esprimono tutto il loro rispetto, la loro vicinanza e il loro affetto nei confronti delle famiglie delle vittime della grande tragedia del 6 aprile e ricordano anche con altrettanto affetto la grande dignità, compostezza e fierezza del popolo aquilano, e anche la straordinaria, generosa vicinanza delle migliaia di volontari

rischiano di diventare delle ricorrenze ad uso interno delle istituzioni se non si ha il coraggio di dire quello che realmente si pensa. Tra le 309 vittime del tragico terremoto vi erano dei bambini, che forse non avevano avuto neppure il tempo di imparare cosa significasse la parola «terremoto»; vi erano degli studenti, che erano lì a L'Aquila per cercare di accaparrare il famoso pezzo di carta che aprisse loro un futuro diverso; vi erano delle madri di famiglia, persone anziane. Il loro ricordo e il dolore delle famiglie, che è tuttora vivo, chiedono al nostro Paese che si faccia chiarezza, che vi sia certezza delle responsabilità, che si arrivi alla verità e si faccia giustizia. Anche al riguardo, le istituzioni possono fare molto, perché saranno necessari procedimenti complessi e lunghi, che potrebbero correre il rischio, alla luce di nuovi provvedimenti legislativi, di cadere

il terremoto del 6 aprile ha delle caratteristiche uniche rispetto a tutti gli altri eventi sismici che hanno colpito il nostro Paese negli ultimi dieci anni. anni. Queste parole assumono tutta la loro veridicità e drammaticità perché L'Aquila in fondo ha subito due terremoti, signor Presidente: il terremoto materiale, che ha raso al suolo una città definita sino a

I miracoli non si fanno, e nessuno di noi abruzzesi ha chiesto che si facessero miracoli, però, signor Presidente (anche al riguardo il Parlamento può fare tanto),

Vi sono ancora 37.000 persone che stanno cercando di tornare nelle proprie case, c'è una zona franca ancora in attesa di trovare attuazione ed una città ancora puntellata e ingabbiata.

cerca di assicurare una vicinanza solidale da parte del Paese e dello Stato nei confronti delle vittime del terremoto, delle loro famiglie e dei superstiti. Credo che la migliore risposta che il Parlamento possa dare sia quella di avviare l'*iter* di questo disegno di legge, rispettando la sovranità del Parlamento, che poi potrà approvarlo, bocciarlo o emendarlo; però la necessità che le istituzioni, soprattutto in questo momento e a partire da questo momento, diano una risposta chiara e definita alle attese, ai bisogni e alle speranze di quelle popolazioni, perché la ricostruzione vera è quella più difficile

Il ricordo commosso va alle vittime del sisma che il 6 aprile di due anni fa ferì a morte la città dell'Aquila, lasciando su questa il suo segno indelebile. Il pensiero corre alle 309 persone - tra loro tanti giovani e bambini - che in quella tragica notte hanno perso la vita, ma va anche alle migliaia di persone che in quel sisma hanno dovuto lasciare le case in macerie e a chi, sotto quelle pietre, ha lasciato la famiglia. Abbiamo tutti negli occhi le tristi immagini di quei giorni, così come restano nella memoria le strade affollate di soccorritori, volontari, forze dell'ordine, gente comune, uniti nell'unico, frenetico obiettivo di riportare alla luce tracce di vita durante le interminabili ore delle ricerche. È straordinario come nei momenti di emergenza e di difficoltà il nostro Paese riesca ad unirsi, profondamente solidale, come una sola persona: lo ripeto, è straordinario. Tutti noi abbiamo seguito con ansia e premura quelle ore e le settimane successive, così come abbiamo accompagnato nelle tendopoli e negli alberghi migliaia di sfollati, documentando le loro vite spezzate e la loro voglia di ricominciare. È seguita poi, subito dopo, l'apprensione per la ricostruzione: siamo stati colti da una sorta di smania di fare tutto in fretta, il prima possibile, per riportare L'Aquila ed i comuni intorno ad una nuova vita che, almeno in parte, ricompensasse quanti ce l'avevano fatta. Eppure, con il passare delle ore, tutto è scemato: solo la disperazione è rimasta intatta.

Ma non è tempo di polemiche, non è giorno di polemica. Constatiamo soltanto che i sogni si sono infranti, che le promesse sono svanite e si sono rivelate inutili. Ebbene, sono convinto che ci sia un solo modo per commemorare degnamente chi non c'è più e per chiedere scusa a quanti, tra i sopravvissuti, fino ad oggi hanno confidato e continuano a confidare nello Stato: bisogna ritrovare la forza di quei primi giorni, recuperando lo spirito di quell'emergenza, che sembra essersi perso nel tempo trascorso. a due anni dal sisma il centro storico dell'Aquila è ancora un deserto sul quale si affacciano simulacri di vecchie case in pezzi e monumenti bellissimi che non ci sono più. Il tessuto sociale ed Il tessuto sociale ed economico di una città giovane e viva sembra essere morto quella notte, e questo deve rappresentare per tutti una conseguenza inaccettabile. Non tolleriamo che questa città torni a vivere soltanto durante la giornata di commemorazione: in 20.000 in piazza questa notte hanno ricordato in una fiaccolata quelle ore di paura. E devono essere proprio queste persone, così come le vittime che commemoriamo oggi, a rappresentare per noi lo stimolo ad andare avanti, a ritrovare quella doverosa voglia di restituire la città e i comuni colpiti dal sisma ai loro abitanti e, soprattutto, occorre fare in modo, con tutti i mezzi e le risorse a nostra disposizione, di restituire la vita a tutti i sopravvissuti, che hanno bisogno della nostra azione immediata.

triste perché in mezzo a quelle vittime vi erano non solo abitanti di altre regioni, ma soprattutto studenti che utilizzavano edifici pubblici e che avrebbero dovuto essere assolutamente protetti.

Oggi dobbiamo dire dei "sì" forti, per una partenza reale e un proseguimento della ricostruzione, per una solidarietà vera, signor Presidente. Questo Parlamento non può approvare

di contenuti e trasferita anche ad altre parti del territorio colpite dal terremoto. Credo anche che il pericolo vero della ricostruzione sia la divisione sociale delle nostre popolazioni, che subiscono spesso ingiustizie e forme di clientelismo fino all'esasperazione. Per questo c'è bisogno di un'assistenza forte, psicologica, che deve durare anni: altrimenti, avremo costruito materialmente una città,

Signor Presidente, penso che sia impossibile per tutti noi cancellare dalla memoria l'angoscia con cui quella mattina del 6 aprile 2009 abbiamo seguito le varie dirette delle emittenti televisive nazionali sul terremoto dell'Aquila; in queste ultime settimane, in seguito al terremoto e al conseguente *tsunami* che ha distrutto il Giappone, penso sia capitato a molti di ricordare quel giorno e il terremoto ha colpito l'Abruzzo. a distanza di due anni esatti da quel tragico evento nel quale, come hanno ricordato i colleghi che mi hanno preceduto, sono morte 309 persone, 1.600 sono rimaste ferite abbiamo avuto quasi 70.000 sfollati, credo sia quanto mai doveroso fermarsi a riflettere, ma soprattutto a ricordare. Questa mattina, alla stessa ora della scossa distruttiva di due anni fa, L'Aquila si è fermata ad ascoltare i 309 rintocchi di campana accompagnati dalla lettura dei nomi delle vittime; alle ore 3,32 di questa mattina 20.000 aquilani hanno atteso in silenzio quell'ora fatale.

la casa, il lavoro e spesso anche la famiglia. È davvero impressionante (mi ha colpito molto) leggere la storia di tutte quelle vite spezzate, così meticolosamente raccolte da una testata locale «Il Centro»: intere famiglie, bambini appena nati, studenti all'inizio della propria carriera.

Ricordiamo la macchina della Protezione civile, i Vigili del fuoco, le Forze armate che hanno saputo gestire l'emergenza con risultati sorprendenti, riconosciuti da tutti anche a livello internazionale. In pochissimi giorni sono riusciti ad allestire 5.000 brande nelle tende e ad ospitare oltre 15.000 persone negli alberghi sulla costa. Nei primi due giorni dopo il terremoto erano attivi sul campo 12.000 soccorritori: pompieri, Forze armate, volontari, vigili urbani, addetti ad elettricità, telefoni e strade. Un impegno veramente immane. Anche qui, sarebbe lungo ricordare le 41 aree di ricovero, i 17 presidi sanitari, tutto quello che è stato messo in campo per dare il primo contributo a quella che era un'emergenza. Ma se all'emergenza è stata data una risposta, diciamo, immediata, ora si tratta di continuare a rispondere alle aspettative della gente. Immagino che tutti abbiamo letto o ascoltato, oggi, le dichiarazioni di Gianni Chiodi, presidente della Regione Abruzzo. Chiodi senza ipocrisia e retorica e con molta sincerità ammesso che: «La ricostruzione all'Aquila e nelle zone colpite dal terremoto dell'aprile 2009 sarà completata non prima di dieci anni». Sempre Chiodi ha poi ricordato che dal 1° febbraio 2010 ad oggi sono rientrate nelle loro case oltre 20.000 persone e che: «Il primo anno è stato dedicato esclusivamente alla gestione dell'emergenza e alla costruzione dei nuovi alloggi. La ricostruzione però inizia con la messa in sicurezza, per la quale nel centro storico dell'Aquila è stato fatto un lavoro imponente». Noi oggi siamo qui a ricordare quelle 309 vittime e per far sentire la nostra vicinanza a chi ha perso tutto, come dicevo prima: la casa, il lavoro, in tanti casi anche i propri cari. Da domani però deve riprendere il nostro lavoro per sanare il più presto possibile questa ferita. Sono certo che tutti noi daremo il nostro contributo e, a nome del mio Gruppo, garantisco tutto il nostro impegno.

Presidente, io non sono disposto a parlare in un'Aula così distratta. Lo faccio sempre, da cinque anni, in qualsiasi momento: ma oggi no.

interminabili rintocchi della campana della Chiesa delle Anime Sante per chi non c'è più hanno risuonato la notte scorsa alle 3,32 all'Aquila, nel silenzio di una città profondamente ferita. Molti di noi erano lì. È stata la notte del ricordo delle 309 vittime di quel terremoto del 6 aprile 2009, a tutti noto. Lo straziante elenco dei 309 nomi e cognomi sembrava non finire mai, e ogni nome è stato una stilettata al cuore dei parenti e degli amici delle vittime. Una veglia composta e silente ha attraversato una città immobile, signor Presidente, distrutta dalla furia di un sisma che durò ben 23 secondi. Quello stesso silenzio avvolge il grande e unico centro storico dell'Aquila e i comuni del cratere da ormai due anni: é il silenzio di tanti che per tenere vivo il ricordo delle vittime hanno raggiunto con una fiaccolata piazza Duomo; quello stesso silenzio in quella stessa piazza che quella notte accolse migliaia di cittadini feriti, spaventati, sgomenti. Tutto intorno, signor Presidente, due anni dopo, solo macerie e tanti puntellamenti. Palazzi sventrati, protesi invano verso il cielo; il grande orologio della piazza, rimasto fermo alle 3,32 di una notte di continue scosse, come le notti precedenti. E poi, la Casa dello studente, o piuttosto quel che rimane di quel simbolo drammatico di una spietata tragedia. Una tragedia, signor Presidente, che - almeno quella - sarebbe stata evitabile se solo la vicina nuova Casa dello studente, a cento passi dalla vecchia interamente venuta giù, fosse stata collaudata e attivata, invece di rimanere vuota, in perenne attesa da ben sette anni, dal 2002. L'Aquila da due anni non sente più i rumori di una vita normale: è sprofondata in un silenzio ancora più immenso. Solo negli occhi di chi ha vissuto in quella città resta il ricordo di un'antica e invidiata bellezza: le sue chiese, scrigni di pittura e scultura, le sue fontane, i suoi palazzi con potenti stemmi gentilizi erano testimonianza dei suoi trascorsi aulici. L'Aquila, città di terremoti, come quello del 2 febbraio 1703 che la rase al suolo, ma da quella catastrofe essa rinacque, ancora più superba, ancora più imponente. Ancora una volta, questi sono gli impegni della politica: chi governa, a qualsiasi livello, deve essere capace di assumersi, solennemente prima e con atti concreti poi, far rinascere L'Aquila e i comuni del cratere dalle macerie erogando loro le risorse finanziarie indispensabili per la messa in sicurezza e per i necessari adeguamenti antisismici della ricostruzione. Far tornare gli abitanti nelle loro case di origine, quelle che permettevano all'Aquila e a quei Comuni di essere vivi, vere perle di bellezze uniche, con i loro borghi stupendi, le loro montagne a un tocco di mano: di essere, insomma, L'Aquila e l'Abruzzo, come li abbiamo conosciuti e come devono tornare ad essere. Gli aquilani attendono, vivi nel ricordo, carichi di una forza d'animo che suscita speranze per il futuro. Un futuro che va pensato già oggi, con maggior concretezza di quanto non si sia già fatto. Nella Giornata nazionale della memoria, che oggi ricorre grazie ad una legge dello Stato che proprio nel Senato, signor Presidente, ha avuto origine per ricordare tutte le vittime delle calamità naturali, il Gruppo del Partito Democratico sceglie di non dare spazio a polemiche, anche se quest'Assemblea sa che purtroppo non sarebbero affatto gratuite, viste le numerose distrazioni e rigidità denunciate in Senato, puntualmente bocciate dalla maggioranza, ma poi tutte accolte dal Governo, a dimostrazione che ponevamo problemi seri e non questioni strumentali. Nel commemorare il terremoto aquilano, oggi ricordiamo innanzitutto le 309 vittime - lo hanno detto tutti - i loro parenti, i loro amici che ancora li piangono, perché tutti loro in quella notte hanno perso gli affetti più cari in quei pochi secondi che hanno distrutto le loro vite e i loro sogni. Scegliamo di ricordare anche - e come potremmo non farlo - le 38.000 persone ancora assistite dallo Stato a causa di quella notte. Il nostro pensiero e la conseguente irrinunciabile nostra azione giunga allora a tutti quei cittadini del cratere che in quella notte hanno perso la propria abitazione, alle 39.000 persone che non vivono più nelle loro case, alle 23.000 persone che sono complessivamente negli insediamenti del progetto C.A.S.E. o nei MAP, ai 2.000 cittadini ancora ospiti tra hotel e caserme.

e 1,7 miliardi di euro, signor Presidente, sono invece pronti per essere spesi, ma giacciono inspiegabilmente in cassaforte. Noi, qui ed oggi, riaffermiamo ad alta voce, convinti e coscienti che le forze politiche non potranno che convenire: ciascuno compia quotidianamente il proprio dovere; ciascuno serva lo Stato, i suoi cittadini, i bisognosi veri con competenza, merito e spirito solidale. Nessuna parola, per quanto sincera e sentita, potrà lenire il profondo dolore di quei cittadini attenuandone l'infinita sofferenza. Al contrario di quanto potrebbe sembrare, oggi i ricordi sono vivi, più che mai, e rendono più amara la consapevolezza dei colpevoli ritardi nel processo di ricostruzione. In conclusione, signor Presidente, alle istituzioni spetta il doveroso compito di non deludere le attese, di testimoniare quanto sia sottile il filo che regge la nostra esistenza e che ci rammenta la nostra innata fragilità. Perché le calamità accadono, inaspettatamente e non lasciano il tempo per l'ultimo saluto, per l'ultimo abbraccio. Allora noi, insieme al Presidente della Repubblica, affermiamo qui oggi, solennemente, e crediamo, insieme a tutti voi, che non vi dimenticheremo mai.

Celebriamo oggi la prima Giornata della memoria dedicata all'Aquila e a tutte le vittime di calamità naturale, con lo spirito di coesione che essa merita e che già quest'Aula ha saputo esprimere, da ultimo in occasione dell'approvazione unanime di emendamenti al decreto milleproroghe presentati dai senatori abruzzesi. Con lo stesso spirito, vorrei esprimere la nostra vicinanza alle popolazioni colpite dal recente cataclisma in Giappone. A loro va tutto il nostro affetto e il nostro più forte senso di solidarietà. Due anni fa lo Stato dimostrò di esserci. L'Italia seppe ritrovarsi unita attorno al dolore dell'Abruzzo, commossa per la solidarietà ed il senso civico dimostrato da tutti quei cittadini, orgogliosa per l'abnegazione e le straordinarie capacità della Protezione civile, dei militari, delle squadre sanitarie, dei Vigili del fuoco, della Croce rossa, di tutte le forze dell'ordine non per ultimi, dei volontari. Oggi è necessario ritrovare e riaffermare quello spirito unitario e costruttivo, superando quel clima di polemiche incrociate e di disinformazione che è sembrato talvolta prendere il sopravvento. Per far questo è necessario dare atto di ciò che il Governo, primo tra tutti il presidente Berlusconi, ha fatto fin dal primo giorno per la comunità aquilana, e che nessuno, in coscienza, può negare. Le fasi della ricostruzione, com'è noto, sono state divise in due parti. La prima è stata gestita direttamente dal Governo, che proprio sapendo della difficoltà e della lunghezza della ricostruzione, in maniera unitaria ha deliberato e legiferato per poter ricostruire il centro storico, e soprattutto per dotare il popolo aquilano,

La seconda fase spetta agli enti locali, i quali - anche questo senza polemica - finalmente stanno facendo i piani di ricostruzione, predisponendo i quali avranno la possibilità - tutti i Comuni del cratere - di rilanciare dal punto di vista sociale ed economico le loro comunità e il loro centro abitato. Per dare concretezza ai piani di ricostruzione sono stati stanziati, fino ad ora, con il decreto Abruzzo più di 14 miliardi. Sono disponibili, come si diceva poc'anzi, in cassa 1,7 miliardi di euro del CIPE un altro miliardo nel 2011. I fondi quindi ci sono. Le promesse sono state mantenute. Si tratta oggi, con il prezioso apporto degli enti, delle comunità locali e di tutti e 57 i Comuni, a cominciare da quello dell'Aquila, di saperli spendere meglio, di investire i denari con efficacia, con chiarezza di obiettivi e con trasparenza. Che la situazione possa evolvere positivamente lo indicano anche altri dati. Si temeva una flessione della popolazione residente, invece il calo demografico ufficiale è stato solo di 700 unità su 75.000 residenti,così come, ad esempio, contenute sono state le defezioni all'università, dove gli iscritti sono passati da 25.000 a 23.000. Queste cifre, per quanto in apparenza fredde, ci danno la speranza, anzi la certezza, che L'Aquila possa e debba rinascere. Occorre spirito di squadra, sinergia e collaborazione da parte di tutti, se vogliamo, tutti insieme, restituire il futuro a questa città. Perché L'Aquila è tutt'altro che morta. È solo ferita. Ha bisogno di ritrovare il proprio slancio vitale. Non serve pertanto a nessuno continuare a paventare complotti o disattenzioni. Non vanno cercati alibi; va invece esaltato il senso di responsabilità. L'Abruzzo continua a proporsi come una Regione laboriosa, che riuscirà a superare la crisi, perché ne ha i mezzi, le risorse e la volontà. Il capitale umano e quello ideale, progettuale e finanziario sono a disposizione. La nostra grande responsabilità sarà quella di saperli amalgamare per farne tesoro in fretta e bene, com'è stato fatto in questi due lunghi ed intensi anni. Possiamo e vogliamo farlo. Ricostruire L'Aquila, le sue mura, i suoi monumenti, le sue scuole, il suo intero tessuto sociale ed economico è ancora una missione prioritaria di questo Governo, di questa maggioranza e di tutte le forze politiche e sociali più responsabili. Con determinazione e capacità lo faremo, rendendo l'onore che merita, nell'anno delle celebrazioni dell'Unità d'Italia, ad un territorio e ad una straordinaria popolazione del nostro amato Paese.

dai dati presentati il 14 marzo dall'associazione Europa Donna, relativi ad una ricerca ISPO, si evince che l'84 per cento del campione intervistato ritiene che di fronte alla malattia bisogna sperare di essere fortunati, poiché non sempre ci si imbatte in strutture e medici competenti. Questo dato assume una declinazione preoccupante anche sul piano dell'appartenenza territoriale: infatti il 57 per cento della popolazione campione concorda sul fatto che chi si ammala al Nord può ritenersi più fortunato di chi si ammala al Centro-Sud. La politica deve cambiare con i fatti questa convinzione; dobbiamo innamorarci di questa causa e percorrere tutte le strade per arrivare a soluzioni positive. Con questo spirito si è conclusa l'indagine conoscitiva sul tumore al seno in Commissione sanità, con voto unanime, lo scorso Da questa volontà nasce la mozione che oggi discutiamo in quest'Aula. Il seno è il simbolo stesso della femminilità, ha in sé valenze emotive forti e racchiude valori che non si possono scindere dall'identità femminile. Per questo è importante che le cure per il tumore al seno preservino il più possibile l'integrità fisica della donna. Prima del 1970, la cultura medica era basata sulla convinzione che più si taglia, più si cura; oggi la filosofia è quella della maggiore conservazione. La battaglia contro il cancro alla mammella è una battaglia sul tempo; è fondamentale dunque che la diagnosi sia il più possibile anticipata, per difendersi e poterlo combattere nelle condizioni più favorevoli. Il carcinoma alla mammella colpisce in Italia una donna su otto, con 40.000 nuovi casi registrati ogni anno; esso rappresenta il tumore più frequente nel sesso femminile e la prima causa di mortalità per tumore nelle donne. L'incidenza di questo tumore ha registrato un aumento negli anni recenti, accompagnato però da una diminuzione della mortalità, grazie alla diagnosi precoce e all'utilizzo di migliori terapie integrate. L'aumento della frequenza del carcinoma mammario deriva principalmente da un drastico cambiamento delle condizioni di vita della donna rispetto alle sue caratteristiche biologiche e fisiologiche, cambiamento legato in gran parte al minor numero di gravidanze, nonché ad una minore durata dell'allattamento. In questa ottica, la cura migliore e più efficace è rappresentata dalla diagnosi precoce, il cui strumento principale e tuttora insostituibile è costituito dalla mammografia. Ciò implica un ruolo attivo delle strutture del Servizio sanitario nazionale, che, attraverso i programmi di *screening*, invitano le donne a sottoporsi all'esame, e un controllo di qualità sulle apparecchiature e la preparazione degli operatori. donne su dieci al Nord dichiarano di essersi sottoposte almeno una volta all'esame mammografico; al Sud, invece, questo accade solo per due donne su dieci. La proporzione delle donne italiane tra i 50 e i 69 anni che, attraverso i programmi di *screening*,

mentre più accentuati sono i dati relativi alla sopravvivenza, con un considerevole 10 per cento in più al Nord rispetto al Sud. Questo è il primo punto su cui intervenire: una revisione globale dei programmi di *screening*. La complessità della malattia cancro della mammella e la sua diffusione hanno fatto si che, negli ultimi anni, si facesse strada la consapevolezza della necessità di una decisa presa di posizione a favore del trattamento multidisciplinare. Con essa si è andato affermando il concetto di *Breast Unit* (Centri di senologia) e di operatori dedicati, intendendosi con il primo termine un luogo di cura che tratta almeno 150 nuovi casi l'anno di carcinoma mammario, e con i secondi un *team* di operatori sanitari che dedicano una parte prevalente del loro lavoro al tumore al seno. Oltre alle figure sopra citate, il Centro di senologia deve inoltre poter disporre, per definizione, di un *team* completo di altri operatori dedicati: alcuni considerati obbligatori, come l'oncologo medico, il radioterapista, il chirurgo plastico, l'anatomo-patologo e il personale infermieristico; altri definiti portatori di valore aggiunto. È proprio tale collegialità e multidisciplinarietà l'elemento portante di un approccio che garantisce alle donne colpite dalla malattia il massimo della competenza e della riflessione, riducendo al minimo il rischio di errore nel procedere terapeutico e allontanando sempre più le donne dal rischio di essere trattate in reparti ospedalieri che non dispongono né di sufficiente esperienza, né di tecnologie adeguate, né di operatori competenti. Vince la squadra, e non il singolo professionista: è questa l'inversione culturale delle *Breast Units*. L'invito che proviene dal Parlamento europeo, e che desideriamo accogliere, è quello di attivare in ogni Stato membro, entro il 2016, un numero adeguato di Centri di senologia con certificazione di qualità: il livello minimo è stato quantificato in almeno una *Breast Unit* certificata ogni 1-2 milioni di abitanti. Un altro capitolo di interesse e di grande importanza è quello dell'ambito farmacologico, con l'introduzione di nuove molecole e farmaci innovativi. Il riconoscimento che si tratta di una patologia eterogenea ha permesso di sintonizzare il trattamento sistemico del tumore mammario con la tipologia delle malattie delle singole pazienti. Infatti, si pone il problema di verificare la qualità intrinseca della cellula neoplastica attraverso lo studio dei marcatori (almeno 50 sono i profili) di proliferazione in modo combinato e lo studio dei bersagli specifici per le molecole farmacologiche adeguate e, di conseguenza, individuare la terapia farmacologica più appropriata. è doveroso chiudere l'analisi di un tema così complesso e delicato citando il ruolo essenziale svolto dall'associazionismo femminile: la spinta che fa emergere il problema, e di conseguenza l'azione, o è di tipo personale perché viene a contatto con la malattia o si manifesta perché ti appassioni ad una battaglia di grande civiltà. L'esperienza americana ne è una riprova. Nel 1993 la suocera di Al Gore, allora Vice Presidente degli Stati Uniti d'America, si ammalò di tumore al seno. Questo fece accendere un grande interesse nello *staff* del Presidente su questa patologia. Nel frattempo, il *pressing* della *lobby* di donne americane fece arrivare più di 500.000 cartoline che chiedevano di iniziare ad investire in ricerca e cura per combattere il tumore al seno. Così fu. Le donne sono state sempre grandi portatrici di grandi battaglie. Il cambiamento che si vuole portare nel campo della prevenzione e cura del tumore al seno non può prescindere da un ruolo attivo della popolazione femminile, perché sono le donne che devono essere le più informate,

di migliorare la qualità dei programmi di *screening* già attivati; di elevare progressivamente il *range* di età delle donne coinvolte nei programmi di *screening*, dagli attuali 50/70 anni alla fascia di età compresa tra i 50 e i 74 anni; di di supportare la sperimentazione di nuove modalità di diagnosi precoce per le donne più giovani (per quanto riguarda la fascia di età 40-50 anni, o almeno con riferimento alla fascia di età 45-50 di introdurre progressivamente per le donne sotto i 40 anni specifici criteri di selezione predittiva basati sui fattori di rischio (gravidanze, allattamento, casi di tumore al seno in parenti di primo grado, obesità), oltre alla mammografia; di promuovere specifici programmi di formazione degli operatori. Con riferimento alle unità multidisciplinari di senologia, si chiede di invitare le Regioni a ridurre l'utilizzo dei centri di senologia che non superano la soglia dei 150 casi trattati per anno richiesti a livello europeo e a promuovere interventi di sostegno, al fine di realizzare nel Paese un numero adeguato di unità di senologia con certificazione di qualità Eusoma, secondo un livello minimo di almeno una *Breast Unit* certificata ogni 1-2 milioni di abitanti; di verificare ed eventualmente disporre una revisione dei relativi DRG, nell'ottica di un DRG di percorso. *(Applausi).*

Per la complessità della malattia e la sua diffusione, il tumore al seno rappresenta una vera a propria patologia sociale in quanto apre nella donna che ne è colpita una vera e propria crisi esistenziale, che è generalmente polarizzata su tutti gli aspetti della vita: il rapporto con il proprio corpo, il significato dato alla sofferenza, alla malattia, alla morte, così come le relazioni familiari, sociali e professionali.

Il secondo punto che pongo all'attenzione del Ministro è legato alla disomogeneità territoriale. La senatrice Bianconi, che prima ha illustrato i vari dati, ha messo in evidenza come sia differente il numero delle

quelle Regioni che sono in ritardo sull'attuazione dei programmi di *screening*, al fine di eliminare queste divergenze ed avere una reale omogeneizzazione, affinché non ci siano anche in questo caso

Desidero sottolineare come l'azione dei parlamentari su un problema così importante sia un segno chiaro di vicinanza ed attenzione a quelli che sono i problemi della gente. Per essere sintetico anch'io, cercando di ottimizzare il tempo, vorrei fare due osservazioni. La prima è che la scienza e la medicina, come lei, signor Ministro, c'insegna, sono in continua evoluzione e vanno avanti. Ogni decisione dipende però da un'attenta valutazione epidemiologica e non da sensazioni. sensazioni. Abbiamo visto come la chirurgia mammaria in questi anni si sia modificata e non ci siano più demolizioni di un tempo; non ci può fermare quindi a quanto già acquisito, anche se molto positivo.

che presenta anche delle alterazioni estetiche molto importanti, e un coinvolgimento, come già si è detto, delle associazioni femminili di volontariato anche nei percorsi decisionali. Sembra che tutto questo si possa concentrare, signor Ministro, nella richiesta di nuovi centri multidisciplinari, almeno uno per Regione, con modelli e sinergie in cui sia presente il chirurgo, l'oncologo, l'anatomopatologo, il chirurgo plastico, il radiologo, il radioterapista, lo psicologo e anche queste associazioni di volontari. In un settore, signor Ministro, in cui spesso si dà molto spazio al privato (quest'ultimo si è preso finora molto spazio), occorre far capire alla gente che non esiste il mago, non esiste il chirurgo straordinario che fa i miracoli, ma può esistere invece una squadra di medici seri che collaborano nel pubblico per rendere più facile e più efficace siamo contrari all'istituzione nell'ambito della scuola di chirurgia della specializzazione di senologia, in quanto un medico non può nascere come senologo; è preferibile, per la difficoltà di questa terapia chirurgica, che a questa si indirizzino già dei chirurghi

perché esse mettono in evidenza significative riflessioni sul tema: per esempio, il fatto che l'aumento della frequenza del carcinoma mammario deriva principalmente dal cambiamento a tutto tondo delle abitudini di vita della donna rispetto alle sue caratteristiche biologiche e fisiologiche, cioè dalla diminuzione del numero di gravidanze per ogni donna e dalla minore durata del periodo di allattamento, sempre che la donna decida di allattare al seno il proprio figlio. Sottolineo la riflessione fatta poc'anzi, perché ritengo fondamentale che le donne abbiano contezza di queste informazioni, in modo tale che esse possano più consapevolmente e responsabilmente operare scelte sia rispetto alla possibilità di procreare di più ed in età più giovane, che sulla rivalutazione dell'importanza dell'allattamento del bambino, soprattutto dal punto di vista psicologico, ottimale per quest'ultimo. Se, da un lato, è stato registrato un significativo aumento del numero di diagnosi di carcinoma mammario, per contro e per fortuna possiamo dire che sono diminuiti i casi di mortalità. Ciò è stato possibile grazie anche alla ricerca medico-scientifica e alla diagnostica precoce, cioè alla possibilità che alle donne viene offerta di sottoporsi periodicamente in tempi non sospetti a visite diagnostiche di controllo, a partecipare dunque a programmi di *screening* anche per donne di giovane La diagnosi precoce, insieme all'utilizzo di migliori terapie di cura, rappresentano lo spartiacque principale tra chi ha la possibilità di guarire e chi non ce la fa. Ecco che i programmi di *screening*, meglio se a tappeto, vista la loro funzione discriminante, devono essere davvero a tappeto e facilmente accessibili. Le donne devono essere informate di quanto sia importante la diagnosi precoce, e devono poter accedere a quelle unità di senologia multidisciplinari previste dalle risoluzioni del Parlamento europeo del 2003 e del 2006. Le *Breast Units*, secondo le caratteristiche dettate dal regolamento europeo, devono garantire un servizio multidisciplinare sia alle donne che dopo l'intervento chirurgico devono sottoporsi alle cure adeguate,

Non basta dunque accompagnare la donna attraverso idonee campagne di informazione sull'importanza della diagnosi precoce; occorre che presso le *Breast Units* sia supportata anche dalla presenza dello psicologo che ha il compito di aiutarla a sostenere lo *screening*, ad impegnarsi a rispettare le periodicità dello stesso

cure e delle numerose visite periodiche, che il carcinoma stesso che, se diagnosticato e curato in tempi corretti, può essere guarito.

che, con l'intento di personalizzare la cura, ricerca, per renderle più evidenti, le differenze esistenti tra uomo, donna, bambino, anziano, sia nelle modalità con cui le patologie si evidenziano che nella risposta alle cure. Il tumore al seno, come è stato detto, è una malattia che colpisce una donna su otto, con 40.000 nuovi casi l'anno, ed è la prima causa di mortalità per tumore nelle donne. Affrontare le problematiche di prevenzione e cura di questo tumore specifico, a mio parere, vuol dire anche entrare nelle strategie del Piano sanitario nazionale 2011-2013 per le patologie oncologiche. A questo proposito, mi auguro che quanto prima siamo messi nelle condizioni di e dare un parere sul nuovo Piano sanitario nazionale, perché, a proposito delle malattie oncologiche, si fa riferimento ad una priorità per cui nell'ambito sanitario occorre incidere con più forza su una serie di patologie che ormai presentano 250.000 nuovi casi l'anno.

il tumore al seno è una delle questioni su cui maggiormente si può forse misurare una frequenza legata anche

di inquinamento dell'aria molto elevati. Se è vero che assistiamo oggi ad una maggior incidenza dei tumori al seno, si registra però anche una riduzione della mortalità. Signor Presidente, colleghi, voglio ricordare, però, che l'Organizzazione mondiale della sanità ha richiamato la nostra attenzione sul fatto che il tasso di mortalità in caso di tumore al seno è ancora superiore al 50

Che cosa fanno le Regioni, a parte inviare una lettera attraverso le ASL e le aziende ospedaliere, per invitare le donne a fare lo *screening*? Ci sono Regioni in cui si va a misurare il livello di fedeltà allo *screening*, che si deve prolungare negli anni, soprattutto per quello che riguarda il tumore al seno?

un trattamento multidisciplinare per migliorare la cura, ma questo tipo di approccio, che molte volte è distante dalla mentalità dei nostri medici, va in qualche modo incoraggiato e incentivato.

nell'ambito del suo piano di cura. Questo non è più accettabile, e laddove queste situazioni ancora esistono - ahimè,

cerchiamo di incidere attraverso questa incentivazione alla creazione di unità multidisciplinari di senologia.

signor Ministro, vorrei pregarla di fare attenzione affinché questo per le Regioni non significhi una concentrazione del personale e una riduzione

entrando direttamente in problematiche davvero importanti per la gente, per le donne e per le famiglie coinvolte da questa gravissima patologia.

e nelle terapie e, infine, nella possibilità di una diagnosi precoce e di un percorso terapeutico uniforme. Questi sono gli elementi fondamentali che ci poniamo con queste mozioni per arrivare a un trattamento sempre più precoce grazie a programmi di *screening*. Non ripeto le puntuali considerazioni fatte dai colleghi

il trattamento, si è parlato di unità di terapia multidisciplinare che prevedono il chirurgo, il radioterapista, il farmacologo, il farmacologo, ma anche l'oncologo, il chirurgo plastico, l'anatomopatologo, nonché personale infermieristico sempre più stimolato e quei portatori di valore aggiunto - come spiega la mozione - quali lo psicologo, il genetista ed il riabilitatore,

paghi e valorizzi la struttura in quanto capace di effettuare nel tempo un *follow-up* che coinvolga la donna nel suo percorso.

di questa patologia femminile, che trova livelli di sopravvivenza sempre maggiori grazie alla capacità organizzativa sempre migliore delle nostre strutture. Dovremmo quindi lavorare per addivenire ad un'uniformità a livello territoriale di questa capacità organizzativa. Ma la strada è tracciata. Permettetemi di aprire una finestra e

cogliere quest'occasione per lanciare anche la volontà di lavorare ancora più nella prevenzione, oltre che della patologia tumorale del seno, così come molto bene è stato fatto con questa indagine conoscitiva, anche di quella

eccezionali che il lavoro fatto sull'epatite B ha dato in questi giorni: mi riferisco alla scomparsa totale di questa patologia nei giovani italiani. È un risultato di cui va dato merito alla programmazione sanitaria di questi ultimi anni. Concludo con una nota ottimista, se me lo permettono i colleghi e il Ministro: in questi giorni stiamo festeggiando i 150 anni dell'Unità d'Italia, che sono stati anche 150 anni di una grande sanità. fu unita, l'aspettativa media di vita degli italiani era di soli 35 anni: oggi, grazie a Dio, le donne italiane hanno, con 85 anni, l'aspettativa di vita italiane hanno, con 85 anni, l'aspettativa di vita più alta di tutto il mondo. Ciò è dovuto certamente alla dieta mediterranea e a tanti fattori ambientali che la nostra bellissima Nazione ha, Nazione ha, ma anche al lavoro silenzioso, oscuro, anonimo, di tantissimi medici, di tantissimi operatori sanitari, di tantissimi infermieri, di tantissimi ricercatori, che in Italia in questi 150 anni hanno lavorato in condizioni di grande disagio e con grande umiltà, ma con straordinarie capacità e professionalità. Credo che questo merito e che in fondo vada riconosciuto anche a tanti politici italiani che in questi anni ci hanno permesso di avere un sistema sanitario all'avanguardia nel mondo, un sistema universalistico

come non mai mettere a massa critica le *Breast Units*; è opportuno ampliare e migliorare il *range* delle

È opportuno, soprattutto - lo cita l'ultima parte della mozione - rendere omogenei i programmi di *screening*; e vorrei ricordare che oggi questo è possibile, perché abbiamo metodi di rilevazione e di controllo. È anche opportuno - ho concluso, ma vorrei lanciare un messaggio importante - creare dei percorsi di continuità assistenziale tra ospedale e territorio. Per questo è opportuno parlare di revisione di DRG, nell'ottica di un DRG di percorso, per creare una reale continuità assistenziale. Questa è una vera novità, onorevoli senatori: non è un qualcosa che è stato espresso in precedenti mozioni. La mozione

sia di puntare l'attenzione su due concetti: diagnosi precoce e terapia ottimale. La diagnosi precoce è necessaria, dato l'aumento della frequenza della patologia, come è stato ribadito da tutti gli onorevoli colleghi, e la terapia ottimale

e come è evidente anche solo dando un'occhiata veloce ai dati e alle statistiche, il tumore al seno è molto più di una patologia grave e rischiosa. Esso rappresenta il principale nemico delle donne, un nemico freddo e spietato, un vero e proprio *serial killer*, che ha come insidia maggiore la non consapevolezza da parte delle vittime dell'attacco letale che stanno subendo. Come è emerso nel corso della specifica indagine conoscitiva svolta presso la Commissione sanità, il tumore al seno è un assassino che non fa grande differenza tra fasce di età. Se per le donne tra i 35 e 45 anni rappresenta la prima causa di morte, con 8.000 decessi annui nel nostro Paese, tale patologia ha tuttavia un'aggressività costante anche nella fascia tra i 50 e i 70 anni e in quella successiva. La pericolosità e la crudeltà del tumore al seno non si esauriscono con ciò che rappresenta la minaccia maggiore, ovvero il forte rischio di morte, ma anche con le conseguenze che, pure in caso di esito positivo delle cure, può lasciare sul corpo, ma soprattutto nell'animo e nella psiche della donna. Avvertire il proprio corpo come estraneo da sé, come un compagno che improvvisamente tradisce e diventa un nemico dal quale doversi difendere, è un processo psicologico inevitabile che si verifica sia negli uomini che nelle donne quando ricevono la notizia di avere un tumore, lieve o grave che sia. Ma questo processo, colleghi, è molto più ampio nel caso del tumore mammario, perché la patologia aggredisce una delle parti più intime e che da sempre connotano l'essenza ed il ruolo quasi ancestrale della donna e del genere femminile. Non è un caso che in tutte le culture del mondo la terra, la fertilità, la vita siano state raffigurate in forme tra loro molto diverse, ma quasi sempre queste figure sono state rappresentate con le mammelle: questa, più di altre parti del corpo, rappresenta la vita, la maternità e la femminilità. Il fatto che il tumore mammario, anche quando viene curato, lasci spesso sul corpo di noi donne il segno del suo passaggio, rappresenta l'elemento che fa di questa patologia un nemico di cui tutte noi donne abbiamo particolarmente paura. Leggendo i dati disponibili, ce n'è uno particolarmente impressionante, ma questa volta in senso positivo. Nonostante il tumore alla mammella nel mondo causi ogni anno 400.000 morti e nonostante in Italia rappresenti la prima causa di morte per donne relativamente giovani, vi è un'altra statistica che indica come la diagnosi precoce assicuri quasi il 100 per cento delle guarigioni per tumori al di sotto dei 2 centimetri di grandezza: la guarigione, in questi casi, dato lo stato precoce in cui la patologia viene aggredita e quindi rimossa, non lascia i gravi effetti deturpanti di cui ho appena parlato. E' un dato che deve farci riflettere, perché rappresenta la chiave di volta per la risoluzione di un problema. Il tumore alla mammella è una patologia grave che mette a rischio la vita delle donne, ma se si effettua una corretta prevenzione, lo scenario si ribalta ed il tumore si trasforma in una patologia certamente preoccupante, ma dalla quale si può guarire. Al di là dei termini tecnici, che lascio alla competenza dei colleghi medici, credo che il concetto più calzante per esprimere il rapporto tra noi donne e questo tipo di patologia sia di considerarla come un "nemico". Ebbene, la migliore difesa da un nemico è anzitutto conoscerlo, diffondendo gli strumenti di conoscenza per individuarlo per tempo. Lo stesso è necessario fare nei confronti del tumore alla mammella, puntando molto sulla prevenzione primaria e secondaria. Il tumore alla mammella è una vera e propria malattia sociale, perché si tratta di una patologia che produce ripercussioni che vanno oltre la sfera della vittima e si allargano ai familiari, agli amici e comportano un costo molto elevato, sia per quanto riguarda le cure (che al Servizio sanitario costano più di 30.000 euro a caso) sia per quanto riguarda l'inabilità che colpisce la persona, la quale, nel periodo della cura, è impossibilitata a svolgere la propria attività lavorativa. L'obiettivo, condiviso da tutti, che si vuole e si deve raggiungere con questo dibattito e con la mozione in discussione è quello di chiedere con forza al Governo in questo caso inteso esclusivamente come istituzione - di fare tutto ciò che è in suo potere per superare le criticità, che ancora si riscontrano nel nostro Paese, nella lotta contro il tumore al seno. In primo luogo, l'informazione, che deve raggiungere tutte le donne italiane ed avvisarle dei rischi che corrono, ma anche del fatto che, con una corretta prevenzione, sia nello stile di vita sia ricorrendo agli indispensabili controlli clinici, la malattia può essere veramente neutralizzata. In secondo luogo, è necessario monitorare ed operare per aumentare la risposta da parte delle donne italiane agli inviti del Servizio sanitario a sottoporsi ai controlli. In questo senso, non è accettabile che il nostro Paese, come hanno dimostrato ancora una volta le statistiche, sia a doppia velocità anche per quanto riguarda la prevenzione del tumore al seno. donne su dieci nel Nord Italia dichiarano di essersi sottoposte almeno una volta all'esame mammografico; al Sud Italia, invece, questo accade solo per due donne su Sono certa che questa condivisione di intenti da parte di tutti i Gruppi, sempre auspicabile quando si tratti di temi di grande e generale rilevanza, darà maggiore valore all'invito che il Senato rivolgerà al Governo. Concludo pertanto, signor Presidente, dichiarando il voto favorevole dell'Italia dei Valori.

Ricordo peraltro che questa è la continuazione di una precedente indagine conoscitiva su tumore al seno e tabagismo, che si era svolta nella XIV legislatura e della quale la senatrice Baio ed io siamo state correlatrici. Lo schema di organizzazione sanitaria che viene proposto da questa mozione per la prevenzione, la diagnosi e la cura del tumore al seno mira a realizzare nel nostro Paese - come d'altra parte auspicato anche dalle mozioni approvate dal Parlamento europeo - un sistema efficace, virtuoso e fortemente umanizzato, che possa accompagnare le donne durante tutto il percorso. Sappiamo che, se la diagnosi viene fatta molto precocemente, le speranze di guarigione e di vita aumentano moltissimo. vorrei semplicemente richiamare il fatto che, se è aumentata la coscienza delle donne e se è cambiata la cultura delle donne, lo dobbiamo moltissimo anche alle associazioni che da anni si occupano di questi temi,

ringraziamento a tutte queste associazioni. In Italia sono circa 1.800 le associazioni che si occupano di salute. Esse sono le vere protagoniste di quella sussidiarietà orizzontale che è indispensabile per creare un cambiamento culturale nei pazienti, ma anche nei medici nel Servizio sanitario in generale; ciò ha permesso di raggiungere, negli anni, risultati positivi per le pazienti. A poco a poco, grazie alla collaborazione tra queste associazioni e molte parlamentari, che hanno costituito una vera e propria *lobby* in questo senso,

importantissimi per la salute delle donne. Per tutti questi motivi, il voto della Lega Nord sarà favorevole. *(PD)*. Signora Presidente, senatrici, senatori, signor Ministro, oggi il Partito Democratico, con molta determinazione e convinzione, dichiara il suo voto favorevole su questa mozione. Il motivo è evidentemente legato al fatto che oggi, nel mondo, circa un milione di donne ogni anno ricevono la diagnosi e la notizia di essere portatrici di un cancro della mammella. Sempre nel nostro pianeta, ogni anno quasi 410.000 donne muoiono di questa terribile malattia. Nel 2010, il cancro della mammella ha rappresentato, come incidenza, il 28 per cento di tutti i nuovi casi di tumore tra le donne. In generale, possiamo dire che una donna su nove viene colpita da questa malattia. In Italia ogni anno vengono diagnosticati 34.500 nuovi casi; i decessi sono circa 11.000. C'è un altro elemento importante che deve essere considerato, e che evidentemente è al centro del concetto di questa mozione, nella costituzione delle *Breast Units*: è il fatto che la nostra popolazione - questa evidentemente è una notizia positiva - arriva sempre più frequentemente all'età anziana. Ma è proprio nell'età più avanzata che il cancro della mammella, come altri tumori, si manifesta di più. Infatti, se a scorporiamo i dati, vediamo che tra il momento della nascita e i 50 anni la possibilità per una donna di essere colpita dal cancro della mammella è del 2 per cento; invece, tra i 60 e i 70 anni arriva quasi al 6 Nel sottolineare l'importanza di questa mozione, vorrei concentrarmi su tre punti. Il primo è quello della diagnosi precoce, delle differenze già sottolineate da altri durante il dibattito questo pomeriggio tra le varie Regioni del nostro Paese. Il Ministro conosce molto bene i dati del Ministero e anche i dati della Commissione d'inchiesta sul Servizio sanitario nazionale. Sappiamo che le discrepanze - questo è un problema che riguarda davvero tutti noi - nel nostro Paese, nello *screening* mammografico, sono enormi. Basti pensare che si va da una estensione dello *screening* che riguarda soltanto il 17 per cento delle donne nella Regione Siciliana a una percentuale che arriva e supera il 90 per cento in Regioni come la Lombardia, l'Emilia-Romagna, la Basilicata e l'Umbria. In termini assoluti, per essere chiari, su 1.000 donne tra i 50 e i 70 anni, oggi in Sicilia vengono sottoposte alla mammografia annuale 59 donne, in Emilia-Romagna 677. È chiaro che c'è una differenza che va colmata. sono i seguenti. È stato pubblicato di recente su «Cancer», una delle riviste scientifiche più autorevoli del pianeta, uno studio eseguito nell'ultimo decennio in Svezia.

i dati di uno studio così vasto dimostrano che si riesce a ridurre la mortalità del 29 per cento. E quindi questo è un altro elemento che va preso in considerazione. avuto come Ministro della salute, ed è anche stato senatore della Repubblica, Umberto Veronesi, che è la persona che nel nostro Paese ha introdotto la quadrantectomia, un intervento importantissimo perché perché riduce quella devastazione anche anatomica dovuta all'intervento di mastectomia che si eseguiva prima di un intervento come la quadrantectomia. Ebbene, purtroppo, nel Paese dove più che in ogni altro si è lavorato scientificamente su questo tema, i dati non sono confortanti. Leggo solo due numeri: nel nostro Paese la quadrantectomia viene utilizzata solo nel 59 per cento delle donne affette da tumore, a Parigi nel 91 per cento, a Boston nel 93 tra una Regione e l'altra, notiamo che in Regioni come la Valle d'Aosta viene utilizzata nel 73 per cento dei casi, in Calabria quasi il 70 per cento delle donne invece viene ancora sottoposta di *routine* all'amputazione della ghiandola mammaria, la mastectomia, perché non vengono eseguite, appunto, le quadrantectomie. Anche questo è un elemento che, come è stato ricordato nell'illustrazione della mozione fatta precedentemente, è evidentemente legato al numero di interventi chirurgici che vengono eseguiti in ogni *Breast Unit*. In conclusione, la diagnosi precoce è davvero importante - è chiaro che

nel fegato o nel polmone, quello che dovremo fare è curare una persona che, di fatto, sarà inguaribile, ma che necessiterà interventi chirurgici molto più pesanti per la sua salute e per il suo equilibrio psicologico, molto più costosi per lo Stato

per quanto più volte oggi ripetuti e apparentemente aridi e noti, i numeri che accompagnano gli aspetti epidemiologici del tumore della mammella ne consentono una lettura funzionale e una valutazione degli interventi che, soprattutto sul versante della prevenzione, intendiamo proporre. proporre. Secondo i dati dell'OMS, circa 332.000 donne dell'Unione europea ricevono ogni anno diagnosi di tumore mammario. In Italia il tumore della mammella rappresenta la prima causa di morte nella fascia fra i 35 e i 50 anni; i dati di prevalenza superano le 450.000 donne, e ogni anno tale patologia è diagnosticata a circa 40.000 donne. Mediamente una donna su 8 sviluppa un carcinoma mammario nel corso della propria vita. Il 5 giugno del 2003 il Parlamento europeo ha approvato all'unanimità una risoluzione della Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità che propone di fare della lotta al cancro al seno una priorità della politica sanitaria degli Stati membri. I due rami del Parlamento, sensibili all'appello del Parlamento europeo, hanno già approvato mozioni sulla lotta al tumore al seno; nel 2005 la Commissione igiene e sanità del Senato

di una nuova e aggiornata indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza sociale, con specifico riguardo al tumore della mammella. Gli obiettivi di questa indagine conoscitiva sono stati i seguenti: fotografare la realtà italiana; verificare la percezione di disuguaglianze nel territorio nazionale; appurare l'accesso alle cure, dopo cinque anni dalla prima indagine conoscitiva sulla situazione in Italia. L'azione più efficace nella lotta contro il tumore al seno è la diagnosi precoce. Alcuni Paesi europei hanno sviluppato piani oncologici volti a ridurre il ritardo diagnostico per migliorare e uniformare il piano di trattamento delle donne con tumore

per cento al Nord, il 73,3 per cento al Centro e soltanto il 27,6 per cento al Sud. La disparità di anticipazione diagnostica dei casi ricade nettamente sulla sopravvivenza a questa malattia, come è ampiamente dimostrato che trattare il tumore della mammella in centri multidisciplinari dedicati aumenta la possibilità di sopravvivenza e soprattutto di guarigione. Secondo la raccomandazione europea, entro il 2016 si dovranno realizzare un numero adeguato di unità di senologia con certificazione di qualità, secondo un livello minimo di almeno una *Breast Unit* certificata ogni 1-2 milioni di abitanti. Pensiamo che le Regioni dovrebbero adottare adeguate misure di dissuasione per i centri che non arrivano a trattare un numero di almeno 150 nuovi casi annui,

con grande convinzione che dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo a questa mozione.

a molti di noi è stato proibito l'accesso ai centri di identificazione ed espulsione (CIE) e ai centri di assistenza ai richiedenti asilo (CARA), in virtù di una circolare emanata dal Ministero dell'interno il 2 aprile scorso. Oggi pomeriggio, mi sono recato a visitare il CIE di Ponte Galeria e non mi è stato permesso di effettuare la visita ispettiva. Ho chiesto di poter visionare la circolare; non mi è stato concesso e mi è stato dato un numero di telefono del prefetto di Roma. Ho chiamato il prefetto e mi è stato detto di chiamare il Gabinetto del Ministro; ho chiamato il Gabinetto del Ministro e mi è stato detto che mi verrà

posto che, almeno da come mi è stato riferito, a qualcuno è comunque concesso l'accesso ai CIE e ai CARA (nella fattispecie, pare - perché appunto ci basiamo su racconti - alle Agenzie specializzate delle Nazioni Unite ACNUR e OIM, ad alcune organizzazioni non governative, come Save the Children), non si capisce come mai ai legislatori, in un momento in cui tra l'altro c'è un'emergenza e gli gli ingressi sono quotidiani, sia proibito (ripeto, stiamo parlando di una prerogativa di tutti i parlamentari: deputati e senatori) l'accesso a tali luoghi, in virtù di una circolare (ripeto ancora una volta, perché sia chiaro il concetto) che non viene fatta conoscere nel suo dettato, ma per la quale ci si deve fidare della parola di un rappresentante della pubblica sicurezza.

distribuito, perché non è possibile andare avanti in questo modo. Dopodiché occorrerà quanto prima affrontare, e nelle Commissioni di merito e magari anche qui in Aula, la questione, perchè solo solo grazie alle visite ispettive nelle carceri, nei CIE e nei CARA si è riusciti, nei giorni scorsi, a portare a conoscenza degli italiani alcuni malfunzionamenti

questa rete di informazioni e di proposte condivise. Basti pensare che abbiamo proposto una distinzione tra prima e seconda accoglienza, la tracciabilità dei minori, la loro identificazione, le procedure giuste. Il nostro Paese quindi avrebbe la possibilità di avvalersi